L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta. Avverte

a nome del Gruppo di Coesione Nazionale, saluto con favore questo importante provvedimento, ringraziando il Governo per il fatto che, nonostante il momento delicato e critico che il Paese sta vivendo in chiave economica e che impone scelte impegnative e di frequente impopolari, trova tempo e capacità per portare avanti questioni che magari per tanti anni da altri Governi sono state lasciate giacere senza alcuna soluzione. È il caso dell'attuazione alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, l'Italia ha promosso importanti convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani, ha posto a fondamento della propria Costituzione il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona ed ha svolto un ruolo importante nella battaglia contro la pena di morte e per l'istituzione della Corte penale internazionale. Manca però fino ad oggi un organismo, indipendente dal punto di vista operativo e finanziario e con adeguato potere d'indagine, che possa vigilare e garantire sul rispetto dei diritti fondamentali della persona umana secondo i criteri fissati dalla risoluzione in questione. Ad oggi, infatti, esistono organismi che rispondono a pieno a tali criteri e sono operanti in 67 Paesi del mondo e in 22 Paesi d'Europa, tra i quali Danimarca, Francia, Germania, Grecia e Irlanda. Altri Altri Paesi, come l'Inghilterra, hanno recentemente riformato il proprio organismo addirittura per renderlo pienamente conforme ai principi di Parigi. Il Ministero degli affari esteri propone a questa Assemblea l'istituzione della «Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani», con il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana. Siamo convintamente a favore dell'istituzione di quest'organo, che avrà anche il compito di predisporre le norme in funzione delle istanze rappresentate dai numerosi comitati dei diritti umani (Comitato per i diritti del fanciullo, Comitato contro la tortura ed altri) operanti presso l'ONU e il Consiglio d'Europa. La Commissione svolgerà anche un ruolo consultivo per il Governo presentando analisi, proposte, pareri e configurandosi come una vera e propria risorsa per l'azione governativa e sarà supportata dal Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, che si configura quale organo consultivo e di indirizzo per la Commissione e rappresentativo della società civile. Insomma, è uno strumento moderno ed efficace per non abbassare la guardia sui diritti fondamentali dell'uomo, che anche in Paesi avanzati come il nostro possono essere messi a repentaglio laddove si creino singole situazioni di mancato rispetto, in particolare nei confronti dei soggetti «meno forti», donne e anziani, dal punto di vista prettamente familiare, e dei cittadini stranieri sul piano lavorativo e sociale in genere. Troppi casi di violenza su base etnica, religiosa, sessuale, eccetera si registrano anche nel nostro Paese. Le forze dell'ordine e la magistratura hanno il compito di reprimerli, ma è fondamentale il lavoro di prevenzione che le forze dell'ordine sono chiamate a svolgere e a cui la Commissione - che ci auguriamo venga approvata al più presto potrà fornire importanti contributi nell'indirizzare gli sforzi lavorativi delle nostre donne e dei nostri uomini a servizio dello Stato. In particolare, l'indipendenza della Commissione sarà elemento fondamentale anche per sgombrare il campo dai molti dubbi che vengono, il più delle volte, surrettiziamente insinuati sull'operato delle forze dell'ordine (vedasi i recenti disordini in Val di Susa o le rinfocolate polemiche per il decennale del G8 genovese). Da convinti donne e uomini di destra quali siamo, ci piace immaginare e sperare che anche grazie all'operato di questa agenzia le forze dell'ordine non potranno più essere oggetto di denigrazioni operate anche attraverso la stampa o comunque mediante canali accessibili a chiunque per il tramite di dati non corretti,

voglio soltanto riprendere oggi alcune delle motivazioni a sostegno del disegno di legge n. 2720. Alla luce di queste argomentazioni, in gran parte espresse nella giornata di ieri, credo che diverse delle posizioni contrarie, che pure ieri sono state manifestate da alcuni di noi, possano essere riviste. Lo faccio molto brevemente. Come più volte è stato sottolineato nella discussione generale di ieri, le norme contenute in questo disegno legge si riferiscono essenzialmente al rispetto di un impegno assunto dal nostro Paese nei confronti della comunità internazionale. E ciò è tanto vero che il testo del disegno di legge mutua quasi integralmente i contenuti della risoluzione 48/134 delle Nazioni Unite. Risoluzione che, voglio ricordare ancora una volta, risale all'ormai lontano 1993. In questi quasi venti anni di "latitanza" (chiamiamola pure così), non solo molti Paesi ci hanno preceduto istituendo le proprie Commissioni nazionali secondo il dettato della risoluzione (e sono stati citati ieri: l'Irlanda, la Germania, il Regno Unito), ma la realtà del mondo si è evoluta in tal misura da rendere ancora più urgente questo provvedimento che, letteralmente, ci mette al passo con la civiltà. L'impegno ad adeguare il nostro ordinamento agli *standard* della comunità internazionale era stato assunto dall'Italia come contropartita all'ingresso nel Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Tutto questo avevo in mente, e soprattutto questo mi stava a cuore nel 2009, quando ho presentato di mia iniziativa un disegno di legge, anche concordato con il Presidente della Commissione per i diritti umani, per l'istituzione dell'Agenzia per la promozione e la protezione dei diritti umani. Per quanto riguarda i giudizi contrari espressi in relazione agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione della Commissione per i diritti umani, faccio notare che, se vogliamo rimanere nel solco tracciato dalla risoluzione ONU, le funzioni attribuite dalla legge alla Commissione non possono essere svolte da altri organi dello Stato già esistenti. La Commissione non può essere accorpata ad altri organismi esistenti in funzione soltanto di un criterio di economie di costo, così come, giustamente, si tende a fare oggi. È necessario che la Commissione si configuri come un'autorità indipendente perché, ripeto, essa deve essere dotata di poteri di inchiesta e investigazione ampi ed incisivi, e deve potere comparire autonomamente dinanzi agli organi giurisdizionali nei casi in cui si ravvisa la violazione dei diritti umani. Deve essere un autorevole e competente punto di riferimento del potere politico, che la deve consultare quando vara leggi e istituzioni che hanno un impatto sui diritti umani. Allo stesso tempo, però, la Commissione deve mantenere la propria indipendenza dal potere politico. E affinché tutto ciò avvenga, a essa devono essere attribuite risorse adeguate al suo funzionamento, così come avviene per le *authority* indipendenti in tutti i Paesi civili del mondo. In poche parole: la Commissione per la promozione e la protezione dei diritti umani non è un nuovo costo della politica! L'*enforcement* dei diritti umani non è un costo della politica! I diritti umani sono la base e il motore della libertà e della democrazia. E lo spirito della risoluzione delle Nazioni Unite recepito da questo disegno di legge è proprio quello di costruire un organismo in "carne e ossa" che promuova i diritti umani, ne verifichi l'attuazione, li difenda, e in concreto li faccia rispettare. Abbiamo finalmente l'occasione di compiere il nostro dovere, quello di un Paese che appartiene a pieno titolo ad una comunità internazionale costruita sulla civiltà, e di presentarci da oggi in poi con le carte in regola dinanzi ad essa.

che in questi due anni è stato molto vicino a me e a tutti i membri della Commissione. il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà con forte convinzione a favore di questo disegno di legge, ma lo farà anche con una forte intenzione critica. approva incondizionatamente l'*incipit* dell'intervento del collega Perduca, che ieri ha cominciato dicendo che vi è violazione dei diritti umani là dove chi dovrebbe farli rispettare non lo fa e ricordava una nota dolente della nostra storia recente, vale a dire la "macelleria messicana" a Genova nel 2001 nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, in cui le forze dell'ordine sono state le forze del disordine. a favore di questo provvedimento perché crediamo, e vogliamo credere con forza, nel sostegno e nella difesa dei diritti umani. I diritti umani vanno presi sul serio, ma per farlo bisogna avere molto ben presente che spesso la società, i meccanismi amministrativi, la politica stessa non li prende sul serio. La rassegna classica dei diritti umani chiama in causa i diritti di di chi è ridotto in schiavitù, delle donne escluse dalle decisioni, dei migranti emarginati, dei carcerati, degli omosessuali, degli zingari, i rom, i sinti, i camminanti o comunque si chiamino. In realtà, l'osservazione della vita ci dice che i diritti umani di queste moltitudini sono tutt'altro che rispettati e garantiti. In Italia indagini giornalistiche serie hanno dimostrato che c'è la riduzione in schiavitù nei lavori agricoli e nella prostituzione. Ci si impossessa di corpi e li si assoggetta senza fine. L'indagine della vita ci dice anche che le due libertà dei classici, la "libertà da", cioè dal bisogno e dalla necessità, e la "libertà di", cioè di scelta e di promuovere le proprie azioni, non sono del tutto salvaguardate. specificato all'articolo 3 della Costituzione, è una meta a cui giungere ma niente affatto un bene garantito per tutti, Costituzione, che dovrebbe garantire la messa in pratica dell'eguaglianza, cioè la progressività dell'imposizione fiscale, è stato rovesciato nel suo contrario: oggi la progressività dell'imposizione fiscale è al contrario, chi ha poco paga tutto e chi ha moltissimo paga poco o quasi niente, se non niente del tutto. È vero che i migranti sono esclusi, maltrattati, sfruttati o supersfruttati e poi gettati via.

ipocrita, ambigua, insinuante, non facilmente individuabile. È vero che i carcerati sono ammassati, vessati a loro vengono sottratti anche i diritti più elementari. Non solo stanno in tre dove dovrebbero stare in uno o in dieci dove dovrebbero stare in tre, ma ultimamente i provvedimenti del Governo hanno sottratto loro la possibilità della rieducazione. Non so se l'Assemblea sa che i docenti delle scuole carcerarie sono stati ridotti a proporzioni minime e che quest'anno molti che si erano impegnati per sostenere gli esami della scuola dell'obbligo non hanno potuto farlo. Gli omosessuali, salvo quelli famosi, importanti, dell'arte e della politica, che vengono allora vezzeggiati, sono spesso irrisi e tenuti in sospetto.

Il collega Livi Bacci ci incoraggiava a tenere sempre presente la duplicità dell'assedio ai diritti umani: il campo nazionale e quello internazionale. avviene regolarmente e quotidianamente nel campo nazionale. Al campo internazionale riservo soltanto un dubbio: è possibile immaginare delle azioni che difendano i diritti umani nel mondo con l'utilizzo di droni, aerei senza pilota, che producono spesso - troppo spesso - carneficine tra le popolazioni civili? C'è una corrispondenza logica e armonica tra il sostegno ai diritti umani e le carneficine involontarie? Noi avremmo votato con piacere un emendamento, ma il presidente Marcenaro mi ha spiegato che esistevano ragioni

ci sono in Italia dei diritti umani fondamentali che vengono conculcati, ed io polemicamente voglio richiamare all'attenzione dell'Assemblea gli ultimi insulti prodotti nei confronti di questi diritti. Il diritto all'informazione e alla conoscenza, che è fondamentale per l'esercizio della consapevolezza democratica, è offeso da una recentissima su una trasmissione televisiva fondamentale, «Report», che conduce indagini sulla realtà, a cui la direzione generale RAI si appresta a togliere la tutela legale. È un'offesa diretta alla possibilità di azione del giornalismo di inchiesta, perché viene ad esso sottratta la tutela legale fondamentale. I cittadini pertanto saranno privati della possibilità di sapere ciò che quella trasmissione di inchiesta riusciva a raccontare, proprio perché il potere ha imposto che le venisse sottratta la tutela legale. E in tema di giustizia, l'ultima cosa cocente, veramente irritante, si verificherà la prossima settimana qui, dove è stato calendarizzato un provvedimento dal titolo ipocrita, che riguarderebbe l'inapplicabilità del rito abbreviato per delitti punibili con l'ergastolo. titolo non c'entra nulla con il vero obiettivo nascosto all'interno di quel provvedimento, che è specificamente l'introduzione del processo lunghissimo tramite l'invenzione della possibilità che un imputato - in particolare il Presidente del Consiglio possa chiamare in causa decine, centinaia di testimoni al fine di rendere impossibile il processo, farlo morire e uscirne fuori per il rotto della cuffia. Questo è un insulto alla giustizia, che dimostra che la maggioranza non ha capito niente dell'ultimo *referendum*, che ha sancito, in modo espressivo e corale, l'insopportabilità per l'opinione pubblica delle leggi *ad personam*.

Presidente, colleghi, la proposta di istituire un organismo nazionale indipendente di promozione e protezione dei diritti umani muove dall'esigenza di dare attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegnava gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli e indipendenti, per la protezione dei diritti umani, dettandone i principi fondanti (i cosiddetti principi di Parigi). L'Italia è uno dei pochi Paesi a non avere dato a tutt'oggi attuazione a quella risoluzione dell'ONU e, pertanto, non ha ancora un'istituzione nazionale, così come proposto dall'ONU. L'attuale Comitato interministeriale dei diritti umani, pur svolgendo un'apprezzabile attività in materia di diritti umani a livello nazionale, non esaurisce tuttavia pienamente le indicazioni della risoluzione dell'ONU, con particolare riferimento ai requisiti di indipendenza e autonomia, ritenuti indispensabili per assolvere a compiti di promozione, e di vigilanza sul godimento, anche in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali così come individuati dalle Convenzioni ONU, dall'Unione europea e tutelati dalla nostra Carta costituzionale. A livello parlamentare è stata dedicata al tema dei diritti umani una grande attenzione. Ricordiamo, in particolare, che in Senato in questa legislatura è stata istituita la Commissione straordinaria sui diritti umani. Si tratta di organismi importantissimi, ma che tuttavia non hanno una durata temporale permanente, ma limitata alla legislatura. Per tali ragioni, è maturata la convinzione di prevedere un'istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, in quanto la loro inosservanza costituisce una delle cause principali dei conflitti e dell'instabilità mondiale. L'azione della politica estera italiana è volta sia a prevenire i conflitti che a ristabilire il rispetto dei diritti umani nei Paesi in cui più gravi e sistematiche sono le violazioni. Il nostro Paese, però, al pari di tutti gli altri Stati, non è immune da rischi di violazione dei diritti umani. Secondo la relazione presentata alcuni giorni fa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, ci troviamo

fondamentali) ha emesso 98 sentenze contro l'Italia, di cui 61 per violazione di almeno un articolo della Convenzione europea, e in 44 casi per eccessiva durata dei processi. A fronte di questi dati, è ormai improcrastinabile creare un'istituzione nazionale indipendente in grado di contribuire a monitorare lo stato dei diritti umani nel mondo in maniera costante. La Commissione deve operare con indipendenza di giudizio e di valutazione, nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria, con i seguenti compiti: monitorare il rispetto dei diritti umani nel nostro Paese; promuovere la cultura dei diritti umani; formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti i diritti umani; contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali. La creazione di questa istituzione appare ancora più necessaria alla luce del ruolo che l'Italia di recente ricopre. Il nostro Paese, infatti, insieme ad altri 14 Paesi, è stato eletto, il 20 maggio scorso, dall'Assemblea Generale dell'ONU nel Consiglio dei diritti umani di Ginevra, per un periodo di tre anni. È un grande impegno per il nostro Paese, che deve farsi portatore di una visione della difesa dei diritti umani, improntata ad alcuni temi prioritari che dovrebbero caratterizzare l'azione della comunità internazionale: la promozione della libertà di religione e di credo e la protezione di tutte le minoranze religiose nel mondo, l'abolizione della pena di morte, l'attenzione verso i diritti delle donne e contro la violenza di genere, l'impegno comune affinché scompaia la pratica delle mutilazioni genitali femminili, femminili, la tutela dei diritti delle persone più vulnerabili e dei minori. Gli impegni internazionali dell'Italia, la sua partecipazione a numerose missioni umanitarie, il suo ruolo di punta nella battaglia contro la pena di morte rendono tale istituzione utile e necessaria. È per questi motivi che, nell'annunciare il voto del Gruppo Unione di Centro e Autonomie, auspico che il lavoro di questa nuova Commissione possa far radicare sempre più la consapevolezza della necessità di una cultura diffusa dei diritti umani per farli diventare anche nel nostro Paese patrimonio di tutti.

lievemente modificato dall'intervento fatto in precedenza dal senatore Pardi, che non esagero nel definire fatto con un po' di arroganza e cattiveria. Ma tant'è! Il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto favorevole al disegno di legge che istituisce questa Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti personali. Nel dibattito svoltosi ieri in discussione generale sono emerse molte sfaccettature che nelle differenze - sale della democrazia - comunque perseguono un obiettivo comune, cioè il bene comune dell'individuo. E questa non è cosa di poco conto. Il ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno dimostrato capacità di sintesi e di determinazione, ad iniziare dal presidente della Commissione dei diritti umani, senatore Marcenaro. Quindi, nel ribadire e rimarcare tutte le considerazioni svolte da me ieri in discussione generale, dichiaro che il voto del Gruppo della Lega Nord sarà favorevole. *(PD)*. Signora Presidente, cari colleghi, naturalmente ringrazio i relatori. La senatrice Incostante e il presidente Vizzini hanno ricordato come stiamo dando adempimento ad una antica risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Hanno ricordato le raccomandazioni pervenute all'Italia

in quello stesso 4 marzo 2011, nel quale il Presidente della Repubblica prendeva la parola con un memorabile discorso davanti al Consiglio dei diritti umani dell'ONU a Ginevra e contribuiva in modo molto significativo al successo dell'Italia, che ha ripreso per la seconda volta nel giugno scorso il seggio al Consiglio dei diritti umani.

luogo, autonomia e indipendenza, che vengono fissate tramite forti regole di incompatibilità non solo con qualsiasi incarico politico ma anche pubblico e attraverso una garanzia di autonomia di gestione delle risorse necessarie per il lavoro luogo, un rapporto con la società civile, e in particolare con il mondo delle associazioni, impegnato sul tema dei diritti umani, le quali comporranno il Consiglio che accompagnerà il lavoro della Commissione e costituiscono una forza fondamentale, come sa chiunque si sia occupato di questo problema. L'Italia è stata attiva nel campo dei diritti umani. state ricordate la questione della pena di morte, le mutilazioni genitali femminili; è stato un lavoro passato ma che continuerà; alla prossima Assemblea Generale dell'ONU, a settembre, l'Italia proseguirà nella propria iniziativa. su questo punto vorrei soffermarmi un momento. Negli anni più recenti, fino alla decisione dell'intervento in Libia, un fatto nuovo, sul quale bisogna riflettere, è stata l'ingerenza umanitaria. Il principio della sovranità nazionale, come si era consolidato nei secoli scorsi, è stato rimesso in discussione: nessuno può fare a casa propria quello che vuole, e la comunità internazionale protegge i diritti umani; nel mondo globale si afferma l'esigenza di forme di regolazione e di governo multinazionali e sovranazionali. si tratta di un processo difficile e lento, a volte contraddittorio, ma questa è la tendenza. La condizione perché l'Italia, come ogni altro Paese, possa portare avanti quest'impegno è che abbia le carte in regola sui diritti umani a casa propria e, in particolare, che rifiuti la pratica del *double standard*, dei due pesi e delle due misure,

una parte della nostra sovranità nazionale per condividerla con altri: la Commissione, infatti, rappresenterà nel nostro Paese e avrà come propria guida non solo il diritto interno, ma anche quello internazionale, quale si forma attraverso i documenti, le sentenze dei diversi *forum* internazionali: delle Nazioni Unite, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte penale internazionale. Alla radice e al cuore dei diritti umani vi è la tutela della dignità delle persone: persone: sappiamo tutti quanto sia importante la libertà; tuttavia, le nostre Costituzioni e le nostre leggi prevedono che della libertà si possa, a certe condizioni, privare una persona. Invece, come ben sapete, non esiste alcuna legge che permetta di privare una persona della propria dignità: neppure chi ha commesso il delitto più orrendo può essere sottoposto a tortura e neppure chi ha fatto le cose più gravi può essere leso nella propria dignità. È molto facile a dirsi, ma molto difficile a farsi. Qui nasce una delle problematiche fondamentali, la formazione dell'opinione pubblica, che è uno dei compiti di questa Commissione. Si tratta di un problema delicato e difficile, perché i diritti umani sono generalmente impopolari, quanto sono spesso i diritti dei "cattivi", o di coloro che sono considerati tali: sono i diritti dei detenuti, sono i diritti degli immigrati irregolari, sono i diritti dei rom, non solo dei "buoni". Informare, combattere i pregiudizi e contribuire alla costruzione di un'opinione pubblica attiva è molto importante. La maggioranza dei Paesi europei dedica risorse importanti, multiple di quelle che decidiamo noi. Osservate invece la sfortuna dei diritti umani: discutiamo di questa legge oggi, in un momento nel quale la costruzione di una nuova Autorità di controllo, come quella che

media europea: se prendessimo come riferimento per i costi di un'organizzazione sui diritti umani la metà della media europea,

che bisognasse mettere il tema dei diritti umani al riparo dallo scontro politico quotidiano, nel quale tutto rischia di essere travolto, compresi i pilastri della nostra casa comune. Abbiamo visto in questi anni principi, che dovrebbero essere comuni, venire prima delle leggi e forse delle stesse Costituzioni; principi che vivono sul confine tra diritto naturale e diritto positivo essere piegati alla propaganda, all'interesse elettorale immediato, alle momentanee convenienze. Con la costituzione dell'*Authority* spero che noi andremo nella direzione opposta. E questo sarà certamente un bene, anche per la qualità del nostro confronto politico. sicuramente la legge avrebbe potuto essere migliore e diversi punti avrebbero potuto avere risposte più avanzate. Abbiamo scelto, consapevolmente, di cominciare, e per questo approviamo convintamente questa legge. Essa è consegnata, per i suoi futuri sviluppi, non solo alla nostra riflessione e alla nostra elaborazione, ma a quella vasta e straordinaria energia della società civile, del volontariato e dell'associazionismo, che con forza l'hanno voluta e richiesta, che da tanto tempo l'aspettavano e ora possono prenderla anche nelle loro mani per farne uno strumento per avanzare nella lotta in difesa dei diritti umani.

nell'Aula del Senato sia un importante provvedimento. Dagli interventi che si sono svolti si è potuta cogliere l'adesione di tutti i Gruppi parlamentari

Council* delle Nazioni Unite e, conseguentemente, l'approvazione di questo provvedimento rafforza quella posizione del nostro Paese. Ma prima di essere un atto normativo, il provvedimento ha una natura ontologica culturale. Per usare l'espressione di Thomas Stearns Eliot, che certamente è anche un filosofo laico, nel suo «Prolegomeni a una definizione di cultura», possiamo dire che la radice dei diritti umani si radica nella religione e nel cristianesimo. Io non condivido la tesi, esplicitata in questa Aula, secondo cui i diritti umani si radicano nell'umanesimo e nella rivoluzione francese. Questi valori sono preesistenti a quegli eventi culturali. Il nostro Paese, di fronte ai diritti umani, ha sempre avuto una grande sensibilità. diceva bene ieri il sottosegretario Caliendo, l'Italia, nel 1948, conformemente anche alla realizzazione di omologhi trattati quali la Carta dei diritti fondamentali e la Carta dei diritti dell'uomo, aveva costituzionalizzato il principio enunciato nell'articolo 2: «L'Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». E pure nella rigidità della Costituzione, noi sappiamo che quello dei diritti umani è un catalogo che rende la nostra Costituzione aperta. aperta. Il senatore Marcenaro diceva che i diritti umani sono i diritti di persone che in questo momento devono essere difese. Io credo che, accanto a questi diritti, vi siano i diritti, anche importanti, delle persone normali, perché il catalogo di questi diritti umani, e lei, presidente Bonino, lo sa, possiamo cominciare a scriverlo con il divieto delle mutilazioni genitali. E lei, presidente Bonino, ha svolto su questa materia un importantissimo ruolo. Il catalogo si allarga anche alla libertà di religione, alla libertà e alla tutela delle donne e dei minori; ma io aggiungo anche la *privacy*, il diritto alla conoscenza e, naturalmente, i diritti delle minoranze. C'è anche da aggiungere, signora Presidente, onorevoli colleghi, che non solo vi è una tutela rafforzata di rango costituzionale, ma vi è anche, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, un ingresso diretto delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo all'interno del nostro ordinamento giuridico. Volevo sottolineare, signora Presidente, onorevoli colleghi, come qui, in questo dibattito che si è svolto, sia stata tralasciata l'importanza che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, assume oggi nel nostro ordinamento giuridico la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non come trattato, ma così com'è stata delineata, cioè secondo l'interpretazione che delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo fornisce il giudice di Strasburgo. Sappiamo che l'interpretazione, quindi il diritto vivente e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è diventata, per effetto del Trattato di Lisbona, norma di diritto interno, che vincola anche l'interpretazione del giudice delle Comunità europee e, nell'ipotesi in cui l'interpretazione di queste norme e questo diritto vivente dovessero confliggere con le norme interne, quindi nel momento in cui si dovesse profilare una antinomia con l'ordinamento interno, vi è il potere dei giudici interni di disapplicare la norma interna. interna. I diritti umani hanno pertanto un ingresso diretto nell'ordinamento giuridico italiano. La realizzazione di questa Commissione determina e caratterizza un impulso culturale e, naturalmente,

determinerà un cambiamento culturale dell'ordinamento giuridico e della cultura del nostro Paese. Certo viene in mente e non ho motivo di nascondere - il dramma che vivono molti detenuti all'interno dei nostri penitenziari. Vorrei ricordare, a questo proposito, la lunga battaglia del Partito radicale di Marco Pannella. Naturalmente questo è un problema che l'Italia deve affrontare, perché, con l'affermazione di questa Commissione, io penso che si potranno anche monitorare quegli spazi di detenzione o di carcerazione che limitano gravemente la dignità dell'uomo, così com'è stato affermato nei precedenti interventi. Credo invece - e non lo dico per una difesa causidica - che sia del tutto improprio l'accostamento che è stato fatto qui

se vi sono state delle violenze o dei fatti di questo genere, voi tutti sapete che vi è una magistratura indipendente, che ha perseguito questi fatti anche in modo duraturo. Ma nessuno può sostenere o immaginare che 400.000 operatori delle forze dell'ordine, che hanno difeso questo Paese dal terrorismo e dalla mafia (ieri li abbiamo ricordati nel sacrificio che è costato la vita al giudice Paolo Paolo Borsellino), nessuno può immaginare che dentro questi corpi della Polizia non vi sia una cultura di protezione e di tutela delle libertà e dei diritti umani, perché questa è la missione principale delle forze di polizia di un Paese democratico, preordinate alla tutela e alla salvaguardia dei diritti, non certo alla loro lesione. Ritengo che ciò sia davvero ingeneroso. Se posso aggiungere un ultimo elemento su quello che è successo a Genova, dico che non vi è stata violazione dei diritti umani, ma, semmai, non vi è stata quella capacità professionale di affrontare situazioni di emergenza, così come i fatti di Genova concorsero a realizzare nella lesione dell'ordine pubblico del nostro Paese.

e rimanda l'Italia ai suoi più alti e immancabili destini di libertà e di difesa estrema dei diritti fondamentali dei cittadini e dei diritti umani. *(Applausi

Le istituzioni sono le prime a non prendere in considerazione la propria legalità, i propri obblighi costituzionali e gli obblighi internazionali che ne derivano. Le istituzioni però, fortunatamente, nella persona del Presidente del Senato, iniziano a manifestare attenzione. La settimana prossima si terrà qui in Senato un importante convegno su quello che è probabilmente il problema dei problemi dal punto di vista della violazione dei diritti umani, ovvero l'amministrazione della giustizia. Non voglio rompere l'unanimità che è stata più volte evocata, e infatti la senatrice Poretti voterà a favore del disegno di legge. Non parteciperò però al voto, anche perché, come ho detto nel mio intervento in discussione generale,

a iniziare l'esame dei numerosi disegni di legge di revisione costituzionale che hanno come oggetto la riduzione del numero dei parlamentari. Non mi risulta che questa sollecitazione in Aula abbia avuto alcun effetto concreto sui lavori della 1a Commissione. Voglio ricordare all'Assemblea, e Commissione. Voglio ricordare all'Assemblea, e naturalmente anche alla Presidenza del Senato, che si tratta di una questione in questo momento di assoluta importanza, non solo per gli equilibri politici del Paese ma anche per lo stesso prestigio del Parlamento. Penso che continuare a ripetere, come la politica italiana sta facendo ormai da anni praticamente quotidianamente e all'unanimità, che si vuole ridurre il numero dei parlamentari e poi non iniziare nemmeno la discussione dei provvedimenti in Commissione

dei provvedimenti che riguardano la riduzione del numero dei parlamentari. *(Applausi

rispetto ad un'esigenza credo avvertita da tutti. A prescindere dalla titolarità dell'iniziativa, se del Parlamento o del Governo, su questo tema della riforma costituzionale (peraltro a tal punto già noto da essere stato oggetto di un *referendum*, che purtroppo non ha avuto un esito particolarmente positivo e significativo, perché una riforma costituzionale in tal senso, seppur all'interno di un quadro più vasto,

perda significato e l'annuncio appaia un rinvio, anziché un impegno. Tant'è, signora Presidente. Ma visto che lei ha ricordato la Conferenza dei Capigruppo,

Mi sembra che in questa direzione si possa e si debba andare per dare credibilità e non strumentalità

lascio alla valutazione dei Gruppi l'opportunità politica di dar luogo ad un dibattito in maniera così estemporanea, e mi si permetta di dire anche platealmente superficiale, rispetto a un tema di questa formidabile portata, sia nella sua oggettività costituzionale sia per i riverberi sull'opinione pubblica. In questo momento, per la parte che mi riguarda, dico soltanto che, trovandomi a disimpegnare momentaneamente

che l'esame di quell'argomento non è mai stato abbandonato e che, anche di concerto e in sinergia con la Commissione affari costituzionali di Montecitorio, si sono tenute molte sedute di lavoro molte audizioni, seguendo un calendario concordato con le Presidenze delle due Commissioni affari costituzionali. Dunque, l'argomento è tutt'altro che passato in seconda o terza linea. Quello che posso dire, per brevità, è che esistono delle proposte di legge (una sarebbe la mia modestissima, che è l'ultima che conta, ma ve ne sono anche altre) che prevedono, soltanto asciuttamente, la diminuzione del numero dei membri di ciascuna delle due Camere. Nulla vieterebbe alla volontà politica dei membri delle due Camere di esaminare asciuttamente e miratamente queste ristrettissime proposte di legge di riforma costituzionale. Ma, perdoni, signora Presidente, mi sembra una precisazione necessaria per noi stessi e per l'opinione pubblica: nessuno ignora, nessun parlamentare di alcun Gruppo, che quasi tutte le proposte di legge di riforma costituzionale che contemplano la diminuzione del numero dei parlamentari la prevedono nel contesto di una riforma del bicameralismo, del sistema complessivamente inteso; dunque, sarebbe assolutamente qui fuor di luogo accusare tutti i Gruppi, tutti i commissari, tutti i proponenti di queste proposte di voler evitare il tema della diminuzione dei parlamentari sol perché lo inseriscono nel quadro di una più complessa riforma istituzionale. Detto questo, concludo dicendo, per la parte che modestissimamente ci riguarda come 1a Commissione, che ove ci sia la volontà politica dei Gruppi e dei partiti di dare impulso prioritario a questo tema non credo che vi sarà alcuna resistenza nelle Commissioni, di Montecitorio e di Palazzo Madama, rispetto

Mi sembra inoltre corretto, senatore Zanda, fare un'altra riflessione. Non possiamo imporre al Parlamento di legiferare o di deliberare sull'onda emotiva creata dai *media*.

costituzionale che volevamo fare noi. Facciamo dunque una riflessione tutti assieme, senza lanciare strali pensando di modificare mille cose, perché la gente

Il mio Gruppo, non anni fa ma due anni e mezzo fa, ha presentato un disegno di legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e per altre modifiche della Carta costituzionale. Oggi non facciamo altro che sollecitare a discutere,

la riforma dell'architettura costituzionale e altre riforme sempre più complicate, che pure abbiamo il dovere di realizzare, non possiamo rinviare tutto alle calende greche. Allora, cominciamo dai punti che ci vedono

Signora Presidente, ritengo utile che il senatore Zanda abbia sollevato in quest'Aula il problema delle urgenze istituzionali e, soprattutto in questo momento critico,

Ciò vale non solo per il numero dei parlamentari, ma soprattutto per la riforma completa delle Camere, inclusa

difendendo nello stesso modo la Presidenza della Commissione, ma sperando che con questa spinta da parte dell'Assemblea effettivamente si possa intraprendere il lavoro. **Discussione

L'articolo 2 (anch'esso rimasto identico) affida all'editore o importatore la determinazione del prezzo da apporre su ciascuna copia e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale non contempli sconti superiori al 15 per cento (tranne che per alcune categorie di libri). Questa è la parte importante del disegno di legge. L'articolo 3 (l'unico modificato dall'altro ramo del Parlamento) fissa la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove disposizioni: dal 1° settembre 2011. A distanza di dodici mesi, dovrà essere elaborata una relazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. Nel testo, come nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, al comma 3 è stato inserito

l'argomento di cui stiamo discutendo e che finalmente giunge alla sua conclusione parlamentare è di enorme delicatezza. di un testo breve, ma molto significativo perché mette un argine a una situazione di deregolamentazione che non ha fatto bene certo alla cultura, all'editoria media e più piccola, alle librerie di medie e piccole dimensioni, quindi al tessuto nervoso della nostra produzione intellettuale, senza nulla togliere ai più grandi gruppi, certo non unici e sufficienti. di norme che già da tempo avrebbero dovuto trovare un'applicazione. Siamo alla terza lettura - il collega Asciutti ha descritto gli articoli con precisione - e finalmente il Parlamento si accinge a varare il testo Mi preme dire, in conclusione di questa doppia introduzione, che il testo che ci accingiamo ad approvare è, naturalmente, a sua volta segnato dal suo tempo. nel lungo percorso che ci ha portato alla terza lettura e - come ci auguriamo - al varo tra qualche minuto, tante cose sono accadute nell'universo

Forse questo testo potrebbe essere persino dedicato a lui, che sarà lieto nella tomba di vedere applicato un pezzo di quel sistema innovativo che proprio il libro

Nessun messaggio e nessun mezzo sono avvicinabili al senso profondo della tavoletta chiamata libro. Ma ora siamo già nell'epoca del libro digitale. Un milione e mezzo di *e-book* venduti entro gennaio 2012, oltre 20 volte il numero di romanzi e saggi digitali acquistati in tutto il 2010. Dunque, dobbiamo offrire questo testo ai nativi digitali, a coloro che sono nati già in questa stagione multimediale, per andare avanti, per immaginare una normativa adeguata al tempo che stiamo vivendo, il tempo digitale. Dunque, che questo testo sia un ammonimento al Parlamento per andare oltre, prima che sia troppo tardi.

tra esigenze diverse che vanno ulteriormente dislocate nel corso della prossima stagione. E quel compromesso positivo andrà spostato più avanti. Il libro è il sintomo della modernità,

signor Sottosegretario, onorevoli senatori, la nostra principale preoccupazione, durante il complesso *iter* di approvazione della legge che oggi si conclude, è stata quella di sostenere le piccole librerie che animano il paesaggio culturale delle nostre città e di rendere possibile la loro coesistenza con le grandi catene di distribuzione, aiutando nel contempo la diffusione della lettura. Per rendere possibile tutto ciò è stato inevitabile agire sulla disciplina del prezzo di vendita e degli sconti e sulla durata delle manifestazioni di promozione; lo abbiamo fatto cercando un punto di intesa tra esigenze diverse. Con questo provvedimento vogliamo sottolineare l'unicità del prodotto libro. Il libro, qualunque libro, è un fatto culturale e come tale va tutelato e non può essere ridotto a mero fatto economico e sottoposto alla pratica dello sconto selvaggio. Per questo pensiamo che sia necessario far sopravvivere le piccole e medie librerie indipendenti, che hanno molto da offrire: innanzitutto la specializzazione e il radicamento sul territorio, un modo per partecipare alla vita di paese e di quartiere e per farlo diventare sempre più un luogo di incontro ed un formidabile polo di attrazione culturale. Analogamente il provvedimento in questione sostiene le piccole e medie case editrici, riequilibrando un mercato sempre più dominato dai grandi editori proprietari di librerie *on line*, di catene di *bookstore*, di fatto un oligopolio in espansione. Da questo punto di vista abbiamo tenuto conto dell'esperienza registrata in altri Paesi, dove l'indefinita e mal regolamentata competizione sul prezzo dei libri si è tradotta in una riduzione del numero delle librerie e talvolta anche in un drastico aumento dei prezzi: è il caso in particolare della Gran Bretagna. Riferimento concreto del nostro provvedimento è stata la legge Lang approvata nel 1981 in Francia. In quel contesto si stabilì il prezzo unico determinato dall'editore, con uno sconto massimo consentito del 5 per cento; tale esperienza ha influenzato altri Paesi europei come il Portogallo, la Germania,

trasmetterà alle Camere una relazione sugli effetti delle nuove disposizioni, una clausola importante che ci consentirà di tornare sulla materia e prevedere eventuali altri correttivi.

intervengo solo per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto. Da tutti gli interventi è emerso con chiarezza che un punto

1a Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.»

in un momento in cui la deregolamentazione in materia di libri ha determinato la chiusura di tante piccole librerie e un'impennata dei prezzi,

a volte, i problemi concreti della nostra società. Così come abbiamo fatto già nel precedente passaggio del provvedimento in Senato, voteremo favorevolmente anche questa volta, felici che finalmente possa diventare legge, provando a risolvere i problemi per i quali esso è stato ideato. In un momento di forte emergenza culturale del nostro Paese, l'Italia dei Valori ritiene importante anche il raggiungimento di questo piccolo traguardo di questo piccolo traguardo della cultura, in luogo delle grandi riforme che in questa legislatura non sono state certamente messe in cantiere. Il presente disegno di legge, già approvato in sede deliberante per due volte dai colleghi della Camera dei deputati, intende disciplinare le modalità con le quali si determina il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e i limiti agli sconti che possono essere praticati rispetto al prezzo già determinato. Così come abbiamo già ribadito in Aula durante la dichiarazione di voto nel precedente passaggio, voglio tuttavia ricordare ancora che di fatto il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta una piccola parte, un articolo, di quello che era il progetto di rivisitazione della materia editoria che lo scorso Governo, dopo una serie di audizioni, si era preoccupato di approntare, ma che non poté portare a compimento a causa della fine anticipata della legislatura. Il provvedimento che approviamo oggi registra la convergenza sia degli editori che dei librai - un fatto importante per noi i quali lo ritengono un compromesso tra le rispettive posizioni riguardo ai modi attraverso cui arrivare alla determinazione del prezzo dei libri. È un provvedimento che trova una giusta sintesi tra il modello tedesco, particolarmente gradito ai venditori piccoli e indipendenti, e il modello inglese (o britannico), più gradito ai grandi editori. Nel modello tedesco, infatti, non è prevista la possibilità di adottare sconti, al contrario che in quello britannico, che prevede il prezzo di vendita libero. Sino ad oggi in Italia si era di fatto realizzata una via di mezzo tra i due modelli, con politiche di promozione sul prezzo e sconti applicati, ma senza che vigesse una disciplina certa al riguardo. l'obiettivo che si è prefisso di raggiungere questo disegno di legge è quello di far individuare liberamente il prezzo di vendita agli editori, prevedendo dei periodi promozionali, realizzabili durante l'anno solare, ai quali i librai potranno non aderire, stabilendo infine un tetto massimo rispetto alla scontistica applicabile. L'Italia dei Valori non può che apprezzare il risultato concreto, quale la normazione di un settore non disciplinato come quello in oggetto: una legge che noi riteniamo buona,

il fine del provvedimento è certamente quello di limitare la concorrenza basata sulle politiche di riduzione dei prezzi tra le diverse librerie, così da consentire la sopravvivenza delle librerie indipendenti che altrimenti sarebbero schiacciate dalle grandi catene. Confermando quindi il principio generale previsto dalla normativa in vigore della soglia massima di sconto del 15 per cento al prezzo di vendita del libro, il provvedimento in discussione prevede alcune fondamentali novità: innanzitutto impedisce alle singole librerie o alle catene di realizzare delle campagne promozionali con la riduzione del prezzo oltre il massimo consentito; fissa poi uno sconto massimo del 15 per cento per le vendite dei libri *on line* e per corrispondenza e infine uno sconto con limite al 20 per cento anche per la vendita dei libri a biblioteche, archivi e musei. Il provvedimento prevede quindi una facoltà per gli editori, a cui la legge attribuisce anche il compito di definire il prezzo del libro, di realizzare campagne promozionali, ma a condizione di non discriminare tra i canali di vendita, consentendo a tutte le librerie di aderire alla stessa campagna promozionale. Ci sono state delle critiche: alcuni piccoli editori hanno criticato proprio tale ultima previsione, sostenendo che la disposizione di fatto consente invece di aggirare gli obiettivi principali della legge. Ciò, a nostro avviso, non corrisponde alla verità, in quanto la norma in oggetto impone all'editore di offrire la promozione a tutti i canali di vendita ed è finalizzata ad evitare la sperequazione tra librerie diverse. Sempre in relazione alla medesima norma, si asserisce poi che essa favorirebbe i grandi editori, gli unici in grado di realizzare delle vere e proprie campagne promozionali a livello nazionale;

la concorrenza in ambito editoriale non è tra due libri diversi, ma tra lo stesso libro venduto in due canali differenti con diverso prezzo. Per questi motivi, a nostro avviso, proporre

tra esigenze opposte, sulla quale il nostro Gruppo esprime appunto parere favorevole. la proposta in esame ha avuto un *iter* piuttosto lungo a causa delle modifiche apportate al Senato in prima lettura, e alla Camera dei deputati in seconda lettura. Essa individua e rappresenta un punto di equilibrio tra le posizioni e gli interessi dei diversi operatori della filiera del libro, editori e librai, grandi e piccoli. Permetterà di tutelare gli interessi dei consumatori, offrendo loro la possibilità di accedere all'acquisto di un libro a prezzi reali più contenuti. Attualmente il settore del libro è in forte crisi. La garanzia di condizioni più agevoli a favore di una platea più vasta di librai e di editori contribuisce sicuramente allo sviluppo del settore librario, tutelando al contempo il pluralismo dell'informazione. Il disegno di legge attribuisce all'editore o all'importatore il diritto di stabilire il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale. Limita al 15 per cento lo sconto praticabile sul prezzo di vendita al consumatore finale, indipendentemente dalle modalità di vendita, riconducendo al potere di determinazione del prezzo di vendita da parte dell'editore o dell'importatore anche la possibilità di realizzare campagne promozionali che, per un periodo non superiore ad un mese, prevedano sconti a vantaggio del consumatore finale, salva la facoltà del rivenditore al dettaglio di non aderire a tali campagne. Può essere praticato uno sconto massimo del 20 per cento. Si escludono dalla disciplina in materia di prezzo di vendita al dettaglio e di sconti alcune categorie particolari di prodotti librari, quali libri per bibliofili, libri d'arte, libri antichi o edizioni esaurite, libri usati, fuori catalogo, pubblicati da almeno 20 mesi, edizioni destinate a rapporti associativi o libri venduti attraverso il commercio elettronico. Si prevede l'ipotesi di prezzo complessivo di collane, collezioni o grandi opere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi, mentre si esclude l'applicazione di norme in materia di vendite promozionali e libri. La legge aiuterà il settore dell'editoria attraverso l'adozione di un modello europeo intermedio simile a quello francese. Un altro aspetto importante è costituito dalla regolamentazione delle campagne promozionali. Non a caso si rileva un vasto consenso sull'iniziativa: il mondo delle librerie, dei librai e delle case editrici è variegato, tra grandi, medie e piccole, con realtà regionali particolari e situazioni diversificate, che necessitano di periodico monitoraggio. L'importante quindi è che le intese raggiunte sugli sconti siano verificate anche dall'autorità *Antitrust*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord all'iniziativa legislativa, che va nella direzione della promozione del libro: il libro, infatti, vuol dire sempre e comunque cultura.

siamo finalmente all'ultima lettura di un provvedimento che ha un generale consenso sia all'interno dell'Aula, sia soprattutto nelle associazioni rappresentative del settore del libro, prime fra tutte l'Associazione italiana degli editori e l'Associazione dei librai italiani. Gli obiettivi dichiarati del provvedimento sono due: il primo è rappresentato dalla difesa di un'offerta culturale diversificata e plurale, da ottenere con la garanzia di un mercato aperto, non dominato e ristretto a pochissimi grandi soggetti, nel quale possano invece rimanere attivi tanti operatori; il secondo è rappresentato dal controllo della dinamica dei prezzi. la nuova disciplina dei prezzi, con due diversi tetti di sconto: uno del 15 per cento, valido per le vendite effettuate da tutti i venditori al dettaglio, dal piccolo libraio alla grande libreria di catena, dal supermercato fino alla libreria multinazionale *on line*; l'altro, del 25

Il duplice tetto agli sconti e la garanzia che le medesime regole e condizioni di gioco varranno per tutti gli operatori dovrebbero infatti permettere di raggiungere il primo dei due obiettivi di cui abbiamo parlato, cioè arrestare l'espulsione dal mercato dei soggetti più deboli e garantire quindi le condizioni per il permanere di una ricca offerta di cultura, svago e informazioni. Queste stesse misure, e in particolare la permanenza nei limiti appena indicati di sconti anche importanti a disposizione, da un lato, dei librai per premiare i clienti più affezionati e, dall'altra, degli editori per promuovere le vendite delle proprie pubblicazioni, dovrebbero consentire poi di raggiungere anche il secondo obiettivo della legge: legge: porre termine ad una guerra combattuta a colpi di sconti sempre più pesanti, il cui risultato ultimo non può essere altro che un continuo innalzamento dei prezzi di copertina, e tutelare i lettori e i consumatori in un momento particolarmente difficile dell'economia nazionale, difendendo il loro potere d'acquisto. Sempre nel merito, vorrei sottolineare e valorizzare il fatto che la legge prevede una verifica degli effetti della nuova normativa a dodici mesi dalla sua entrata in vigore: si tratta di una previsione che si dovrebbe applicare a qualsiasi nuova legge, ma in questo caso, trattandosi di un provvedimento che modifica le regole del gioco di un mercato, è ancora più importante. Dichiaro dunque il nostro voto favorevole ad una legge equilibrata, frutto del lavoro di ascolto di tutti gli operatori del settore

Levi. Ogni iniziativa di sostegno alla lettura, in un Paese, come l'Italia, che condivide con la Grecia il triste primato del più basso livello di consumi culturali, rappresenta comunque un obiettivo importante. importante. In conclusione, mi sento di dire che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che, se non per i suoi tempi di esame, certo per il merito e per il metodo costituisce un esempio di buona legislazione e di dialogo proficuo tra le forze politiche.

Signora Presidente, oggi ci troviamo a discutere e a votare un provvedimento sul prezzo dei libri: quindi parleremo di soldi e di cultura, due concetti che sembrano assai distanti, ma che invece ai giorni nostri sono strettamente in relazione. Voglio citare al riguardo una breve constatazione del celebre scrittore Erri De Luca, il quale, nel breve saggio intitolato «Tentativi di scoraggiamento (a darsi alla scrittura)», asserisce che «è civile il tempo in cui *carmina dant panem*». un assunto che vale ben poco per gli scrittori, in quanto ai giorni nostri sono purtroppo uno sparuto gruppo coloro che riescono a sostentarsi soltanto grazie alla vendita delle proprie opere. Eppure, è una frase che ben può valere per quelle piccole librerie e per quei meravigliosi librai che ancora oggi riescono a resistere con i loro minuti negozi nei centri storici delle piccole e grandi città nonostante la vasta proliferazione di megalibrerie e centri commerciali. Un tempo eravamo adusi ad acquistare le copie dei nostri scrittori preferiti nelle numerosissime piccole librerie. Per fortuna, ancora non sono scomparse del tutto, e magari anche voi avevate un vostro libraio di fiducia che vi consigliava un libro da leggere. Bei tempi, quelli in cui, al nostro passaggio all'esterno della vetrina della libreria, il nostro libraio ci avvisava di un nuovo arrivo. Comunque, parlandone più in concreto, con questo provvedimento si intende fissare un tetto massimo allo sconto applicabile ai libri: che il prezzo sia quindi scontabile fino al 15 salvo casi eccezionali per particolari campagne promozionali, che non potranno durare comunque più di un mese e non nel periodo natalizio. Si potrebbe pensare che con questo provvedimento intenderemmo limitare la libera concorrenza tra le librerie. Non è così. Questo è semplicemente un responsabilissimo rimedio che mira a tenere viva e capillare la vendita di materiale culturale nel nostro Paese. È questa legge un modo per salvaguardare le piccole librerie dal potere della grande distribuzione, che più agevolmente ha la facoltà di effettuare sconti e riduzioni grazie a un più importante potere di acquisto (senza comunque demonizzare le grandi librerie che svolgono, anzi, un compito fondamentale, essendo divenute nel tempo dei veri e propri centri di aggregazione presso cui è possibile incontrarsi e promuovere importanti attività culturali). Le librerie, in fondo, non sono soltanto dei luoghi presso cui è possibile acquistare dei libri. In un senso più ampio, altro non sono che dei centri culturali. L'Italia è il Paese e la culla della cultura per eccellenza, e meglio riusciremo a preservare e promuovere la capillarità di questi nostri centri culturali, meglio sapremo conservare il buon nome della nostra identità. Con questo provvedimento riusciremo a tenere in vita la struttura vitale dei centri di diffusione culturale delle nostre città, sperando che, anche grazie a questo accorgimento, si riuscirà a incentivare più persone al piacere della lettura. in futuro, spero presto, potremo discutere anche di iniziative e provvedimenti che possano incentivare i nostri cittadini, soprattutto i giovani, alla lettura. La discussione odierna può infatti essere un'ottima occasione per svolgere una breve riflessione. Molto spesso siamo così occupati occupati a salvaguardare la nostra immagine di Paese a vocazione culturale presso l'estero, al fine di favorire l'*appeal* turistico del nostro Paese, che quasi dimentichiamo come tenere viva questa tensione culturale presso i nostri stessi concittadini. Se non faremo ciò, disperderemo un fondamentale patrimonio del nostro essere italiani. Cultura, in fondo, non è soltanto quella che si insegna nelle scuole. Forse, sono ancora più importanti le esperienze che è possibile formarsi all'esterno degli istituti scolastici, magari proprio attraverso letture personali che favoriscono quella sorta di autoapprendimento così prezioso per ogni individuo. Colgo l'occasione di questa discussione per invitare tutti a far proposte in tal senso e a discuterne in quest'Aula prossimamente. Per concludere, il disegno di legge che oggi votiamo è certamente un mezzo utile per meglio favorire la diffusione di cultura nel nostro Paese. È un piccolo grande passo per salvaguardare le piccole grandi aziende, così come gli stessi fruitori. Per questi motivi, nel ringraziare tutti coloro che hanno discusso e migliorato questo testo, sia in quest'Aula che alla Camera dei deputati e in Commissione,

Proprio in questi giorni, in cui si fa un gran parlare di casta accusando la casta della politica, questo provvedimento ci rientra a pieno titolo. Stavolta si parla di un'altra casta, quella dell'editoria. Ancora una volta siamo qui a sottolineare che questo è un provvedimento un provvedimento corporativo e protezionista, che vede il mercato come un qualcosa di pericoloso, come una giungla non da regolamentare e da disciplinare, ma da cui scappare a gambe levate. Questo provvedimento dovrebbe invogliare

l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga di missioni internazionali avrà inizio nella seduta pomeridiana di oggi.

Presidente, io lamentavo il fatto che tra i collaboratori della Cassa nazionale dei ragionieri che, dopo aver investito in titoli tossici, doveva mettere sul mercato gli immobili e mettere alcuni inquilini in mezzo alla strada, c'era l'architetto Maurizio Mazzotta. Questo signore era una vecchia conoscenza della giustizia, collaboratore di Francesco e già condannato a otto anni di reclusione nell'ambito del crac del vecchio Banco Ambrosiano. Ora, si dà il caso che il presidente di questa cassa, Paolo Saltarelli, scriva una lettera indirizzata al dottor Luigi Bisignani, piazza Colonna 370, 00186 Roma: «Caro Luigi, è con grande gioia che ti scrivo per ringraziarti a nome di tutto il Consiglio, per aver sbloccato la situazione dismissione immobiliare con gli amici del Ministero. In questo Paese le leggi sembrano fatte apposta per bloccare le nostre attività ma noi non ci arrendiamo. Ti aspetto a Milano a presto». signora Presidente, noi come politica siamo sotto il ricatto dei faccendieri e di coloro che si vendono le nomine della P4. Ci sono persone ed inquilini che andranno in mezzo a una strada per i cattivi investimenti fatti anche su titoli